Comunico che, in data 4 giugno 2021, l'onorevole Gennaro Migliore, componente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, è stato eletto Presidente dell'Assemblea stessa. All'onorevole Migliore vanno le più vive congratulazioni, unitamente al sentito augurio di buon lavoro. ln sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusura durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto di due decreti-legge, il decreto-legge n. 56 del 2021 e il decreto-legge n. 65 del 2021, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti. Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e un allegato. L'articolo 1 riguarda la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. L'articolo 2-*bis,* introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni sulla disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. L'articolo 2-*ter* impegna il Ministero ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che assicuri il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, lo svolgimento delle visite da parte dei familiari ovvero l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare. L'articolo 2-*quater* prevede che alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali, munite delle certificazioni verdi Covid-19, siano consentite uscite temporanee. L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione la possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla. L'articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli Il nuovo articolo 4-*bis* dispone che in zona gialla possano svolgersi, anche nei festivi e prefestivi, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali, gallerie, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili. L'articolo 5 detta disposizioni sullo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi. Il nuovo

7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere dal 15 giugno e di convegni e congressi dal 1° luglio. L'articolo 8 prevede la riapertura in zona gialla delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento. L'articolo 8-*bis* dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del terzo settore e la ripresa, in zona gialla, delle feste. Il nuovo articolo 8-*ter* consente, in zona gialla, l'attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi Covid-19. L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. Il nuovo articolo 10-*bis* modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali. L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio il termine delle disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al decreto-legge a parte alcune eccezioni espressamente indicate. I nuovi articoli da 11-*bis* a 11-*duodecies* recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, quella al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento d'identità con scadenza 31 gennaio 2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione in scadenza sino alla medesima data. L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico. Il nuovo articolo 12-*bis* norma lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su su strada di merci e viaggiatori, in modo che siano sempre consentite. Il nuovo articolo 12-*ter* consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto *voucher* taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali. L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria. L'articolo 13-*bis* reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

un semplice atto amministrativo, che però ha bloccato un Paese. Abbiamo anche letto - vero o falso che sia - che addirittura c'era un'ideologia

in quest'Aula alcuni colleghi ci hanno attaccato sulla gestione dell'ospedale di Milano, che oggi è stato il fulcro e ha aiutato la situazione di quella Per fortuna ci siamo anche noi, oggi, in questo Governo, che parla di ripresa delle attività economiche. Ben venga: parliamo solo di ripresa delle attività economiche e speriamo che ci sia comunque il blocco dell'attività dell'immigrazione clandestina, che oggi sta arrivando con forza del nostro Paese. Grazie e buon lavoro a tutti.

dopo i diciotto mesi più difficili della storia recente, possiamo guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo e, se possiamo farlo, è grazie alla prudenza e al rigore con cui è stata affrontata la fase più ardua della pandemia. Il rischio ragionato con cui è stata gestita l'emergenza degli ultimi mesi sta dando i suoi frutti e ne va dato atto a chi, come il Presidente del Consiglio e il Ministro della salute, ha deciso di agire con lungimiranza, in base all'evoluzione del quadro epidemiologico, senza pericolose corse in avanti, per inseguire i sondaggi. Per noi del Partito Democratico questa è stata una strategia ottima e infatti l'abbiamo sostenuta fin dall'inizio, perché ci ha consentito di riaprire progressivamente le attività, anche in ragione dell'accelerazione della campagna vaccinale, senza correre il rischio di richiudere. Aprire e poi richiudere sarebbe stato infatti un dramma, che avrebbe messo in ginocchio definitivamente il Paese. Non abbiamo ceduto alla facile propaganda e agli *slogan* e credo che questa serietà ci abbia premiato. In questo senso siamo soddisfatti di aver sostenuto l'azione del *Premier*, l'agenda Draghi, una strategia che ha cercato sempre di tenere saldamente unite la salute e la sicurezza dei cittadini, con il rilancio dell'economia, che infatti mostra chiari e inequivocabili segni di ripresa. Va dato atto anche al grande senso di responsabilità degli italiani e alla fiducia mostrata, se questa ripresa oggi è possibile. *(Brusìo).* Scusi, e il rispetto delle regole sono stati elementi decisivi per permettere la riapertura del Paese e il progressivo allentamento della limitazione negli spostamenti. deputati ha inoltre apportato delle utili modifiche in sede di discussione parlamentare e questo è un elemento importante, che tengo a sottolineare, perché la centralità del Parlamento non va mai dimenticata e va anzi valorizzata. al nostro esame lo stato di emergenza viene prorogato, con una scansione delle aperture che consente di continuare a gestire la crisi epidemica e, contemporaneamente, di far ripartire le attività economiche, sociali, culturali ed educative. Si tornano ad aprire gradualmente le attività economiche, la ristorazione, le attività sportive, i luoghi di socialità, i centri termali, tutte attività che in questi mesi hanno cercato di tenersi a galla, in qualche modo, grazie ai ristori e ai sostegni precedentemente varati, ma che aspettavano con ansia la riapertura e il ritorno al lavoro. I ristoratori hanno potuto finalmente riprendere la loro attività, dapprima all'aperto e ora anche negli spazi interni. Penso poi in particolare alla nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con il protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid-19, oppure all'introduzione, nelle attività dei servizi educativi, dei corsi di formazione specifici. temi che mi stanno particolarmente a cuore, il primo perché riguarda il difficile mantenimento delle relazioni familiari anche in presenza di contagi o di malattie croniche e il secondo perché concerne la qualità delle relazioni educative. anche ricordare la grande, grandissima importanza dell'apertura al pubblico dei musei e degli istituti di cultura, per esempio limitando la necessità di prenotazione preventiva nei giorni festivi e di sabato. Sappiamo bene quanto abbia sofferto il mondo della cultura e dello spettacolo in questi lunghissimi mesi e quanto abbia bisogno di ripartire e di riaprire. Stiamo tornando finalmente alla normalità, alla vita, al lavoro, alle relazioni che costituiscono una parte fondamentale delle nostre esistenze e lo stiamo facendo attraverso il rigore e il buonsenso. Bisogna ribadirlo con forza: senza il rischio ragionato, inseguendo invece le sirene del consenso immediato, probabilmente non saremmo qui. È proprio grazie al rigore e al buonsenso che le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno potuto completare, per esempio, l'anno scolastico in presenza, almeno alla conclusione, dopo mesi di didattica a distanza e di perdita della quotidiana relazione con le compagne e i compagni di classe. Si tratta di una vittoria, perché tutti noi sappiamo la portata del dramma che hanno vissuto molti bambini e adolescenti privati della scuola in presenza, delle relazioni sociali e umane indispensabili per la loro crescita educativa equilibrata. La crisi sanitaria sulle loro vite è stata come una crepa su una fragile diga, ha aperto uno squarcio che ha sconvolto il mondo delle relazioni e le identità in costruzione. In particolare, gli adolescenti sono stati alle prese con evidenti problemi emotivo-relazionali e sociali e sociali caratterizzati da incertezza, ansia, paura, dolore preoccupazione, ma anche disorientamento, apatia, paura del futuro. Non possiamo ignorare, quindi, la necessaria ripartenza anche in merito a questo fronte delle riaperture. Nel pieno dello sviluppo cognitivo comportamentale, ma anche sociale e pedagogico, in quella complessa fase di passaggio che porta alla vita adulta, molti giovani hanno perso punti di riferimento, rapporti solidi a scuola o in famiglia, legami educativi certi. Un diffuso analfabetismo dei sentimenti, vacillanti tra mille incertezze esistenziali, che spesso non hanno trovato parole per essere dette, ha ulteriormente indebolito il sistema delle regole e, dunque, ha prodotto chiusura su chiusura dentro i mondi virtuali, che tanto male possono fare, se non mediati o se utilizzati in modo non consapevole, acuendo dipendenza e isolamento. Di queste criticità ci stiamo già cominciando ad occupare tramite alcuni ordini del giorno o risoluzioni già approvati, ma serviranno interventi psicologici e pedagogici sempre più mirati e significativi e, soprattutto, serviranno le aperture. La medesima attenzione riguarda l'ambito sanitario, per facilitare ad esempio gli spostamenti all'interno dell'Unione europea o contribuire alla ripresa economica anche con il cosiddetto *green pass*, ma, soprattutto, consentire la possibilità di accesso come visitatori ad alcune strutture di ricovero e di assistenza. Siamo dunque tutti consapevoli che i cittadini hanno bisogno di un ritorno alla mobilità, alle relazioni sociali, alla vita per ciò che è sempre stata. Per questo le istituzioni devono essere molto attente nel comunicare le scelte che si compiono in materia sanitaria, perché non bisogna creare diffidenza o paura, ma accompagnare i cittadini in questa fase complicata per tutti e i nostri concittadini stanno dimostrando di avere una grande responsabilità, fiducia e voglia di ripartire. Nel frattempo, è importante ricordare che è necessario tenere alta la guardia, perché il nemico non è ancora stato battuto e quindi è indispensabile continuare ad agire, in ragione di un rischio calcolato, che tenga conto di ogni variabile, a partire proprio dal quadro epidemiologico. In conclusione, dobbiamo marciare insieme uniti. Quello attuale è un Governo di larghissima maggioranza, nato su impulso del nostro autorevole Presidente della Repubblica. È un Governo che deve fronteggiare la peggiore crisi, sanitaria, sociale ed economica dal Dopoguerra a oggi. Per questo motivo serve che tutti remino nella stessa direzione. Siamo convinti che l'agenda del Governo Draghi per la riapertura, la ripartenza e il rilancio del Paese sia quella giusta, allo stato attuale delle conoscenze e delle possibilità,

È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

pass.* A noi non sembra corretto che chi non può o non vuole vaccinarsi sia svantaggiato rispetto a chi invece ha deciso di farlo.

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Riteniamo che questi emendamenti siano molto importanti, perché non è giusto che chi si vaccina possa farlo gratuitamente mentre per chi, invece, decide di non farlo,

si è espresso in maniera contraddittoria sulla prescrizione delle somministrazioni di alcune tipologie di vaccini, come per esempio AstraZeneca. Sappiamo tutti che vaccino è estremamente contestato: inizialmente è stato prescritto a chi aveva meno di sessant'anni. Successivamente, dopo i primi decessi, si è pensato di

sa che tipo di vaccini consigliare a quale fascia d'età e a quale tipologia di cittadini, e ha dimostrato grande incertezza (e d'altra parte non poteva che essere così, dato che questi vaccini sono ancora in fase di sperimentazione), ancora di più ci sembra doveroso prendere atto che hanno diritto ad ad essere trattati come gli altri tutti i cittadini che decidono di non sottoporsi alla vaccinazione, perché anche questa è una scelta legittima, è una scelta riconosciuta dal nostro ordinamento e quindi deve avvenire con pari opportunità. Ecco perché

accolgano i nostri emendamenti che si limitano ad adeguarsi al dettato costituzionale, quello sempre calpestato e vilipeso da quest'Aula, ma anche dallo stesso Governo che impone limitazioni senza offrire alternative che sono nei diritti di tutti i cittadini. Anche l'articolo 16 della nostra Carta costituzionale prevede. Ma poi c'è la libertà di associazione e di manifestazione: sono tutte libertà che vengono negate a chi non ha la possibilità o non ha la volontà e l'intenzione di vaccinarsi. Anche la scelta libera del soggetto che

passato il vaglio della Camera dei deputati) che rappresenta un passaggio significativo e decisamente innovativo

con i decreti-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Tale pratica certamente depauperava quello che a noi parlamentari interessa, e cioè la centralità del Parlamento, la funzione stessa che noi parlamentari dobbiamo svolgere, l'attività legislativa. Di fatto, noi siamo stati defraudati per troppo tempo, per troppi mesi, con lo spauracchio della pandemia e della necessità di fare in fretta, della facoltà di lavorare secondo gli strumenti che ci ha conferito la nostra Carta costituzionale, ai sensi dell'articolo 77 della nostra Costituzione. Noi ne siamo stati defraudati.

secondarie ma che, in questo anno terribile, sono state invece fondamentali. Hanno quindi ripreso vita, in termini di funzione legislativa, la disciplina delle attività scolastiche; l'attività dei servizi di ristorazione; la disciplina degli spettacoli aperti al pubblico e anche degli eventi sportivi; la disciplina delle palestre, delle piscine e degli sport di squadra; la disciplina delle fiere, dei convegni, dei congressi

Il secondo aspetto che rappresenta - a mio giudizio - forse quello politicamente più significativo - cari colleghi, e soprattutto cari colleghi di Forza Italia - è che, per la prima volta, il Presidente

che si assumeva un rischio ragionato nell'affrontare le riaperture anche prima di quanto affermavano alcuni cosiddetti virologi che imperversavano nelle televisioni va detto, perché è stata la prima volta in cui - a mio giudizio - da quando è iniziata la pandemia, si è verificato il cosiddetto vero e proprio cambio di passo.

hanno dato ragione quella decisione dalla quale poi sono discesi questi decreti-legge accordati.

non solo la dignità, ma anche quel valore garantito dalla Costituzione e a cui un partito come il nostro, Forza Italia, tiene più di qualunque altro: la libertà

in pochi giorni tutti dimentichino quello che è accaduto soltanto ieri o l'altro ieri. Invece noi dobbiamo avere ben chiara l'idea che con il Governo in

tutta Forza Italia siamo orgogliosi di avere finalmente un Capo del Governo che si assume certe responsabilità anche rispetto a temi scottanti della politica internazionale Non ci imbarazza dire esattamente come stanno le cose. Concludo citando alcune parole della collega Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia la quale alla Camera dei deputati ha ricordato che, con il decreto-legge in esame, molte cose sono mutate in positivo e che la libertà è un valore costituzionalmente garantito insieme ad altri valori importanti, come il lavoro e la libera iniziativa. Grazie al decreto-legge in esame, che anticipa le riaperture rispetto alle date previste, siamo riusciti ad ottenere un importante risultato e a garantire le attività in tutta sicurezza, adottando tutti quei protocolli che consentono di tutelare anche quell'altro bene importante garantito dalla Costituzione, e cioè la salute. Ho voluto ricordare le parole della collega, perché ritengo abbia detto esattamente quel che andava affermato nei confronti di un provvedimento del genere. Io vi ringrazio e ringrazio ancora Forza Italia che ha avuto il coraggio e la forza di sostenere Mario Draghi come Presidente del Consiglio dei ministri. Ha fatto molto bene!

messi in atto dal momento in cui il nostro cielo si è oscurato. Forse era dal Dopoguerra che non avevamo un periodo

ne ha sentito parlare dai suoi nonni, dai suoi parenti, ma nessuno l'ha potuta vivere. Invece, noi ci siamo trovati in una situazione

Senatrice, con tutto il rispetto, io la ascolto e devo anche richiamarla a un linguaggio consono all'Assemblea.

Benissimo, continuo a parlare di questo provvedimento che chiude un elenco di altri provvedimenti che ci hanno messo nella condizione, purtroppo, di far emergere non solo delle difficoltà sotto il profilo sanitario sul come affrontare una malattia sconosciuta. Questo ci è capitato: ci sono stati molti morti e molti medici morti. Abbiamo dovuto rincorrere all'inverosimile con ogni mezzo e tante volte i mezzi sono stati inefficaci. Ci siamo trovati ripeto - dal Dopoguerra in una condizione cui non eravamo preparati, soprattutto perché, se da una bomba, bene o male, pur nel disastro causato dalle guerre e dalle violenze perpetrate, ci si poteva nascondere,

però, il punto fondamentale di come si riapre. Ci sono state diverse colorazioni a seconda della gravità della situazione regionale e locale della malattia, ma nelle

Tanti hanno smesso di andare a scuola perché c'è stato un cambiamento radicale che forse viene portato troppo poco all'attenzione. Ci sono tante proroghe nel provvedimento. Ce ne sono state tante.

non dovrete preoccuparvi tra sei mesi di andare all'Agenzia a pagare, visto che non avete guadagnato. Ci accolliamo noi i debiti e, quando vi riprenderete la vostra vita, come si sta cercando di fare adesso,

oppure onniscienti, non saremmo neanche in quest'Aula, perché faremmo tutto da soli e non avremmo bisogno di stare delle ore a discutere anche sulle piccole virgole. Il virus è lì e vedremo che fine farà

Dobbiamo ricordare che l'esperienza che abbiamo vissuto è stata pesante, e che alcuni di noi hanno vissuto sulla propria pelle, me compresa.

la lotta alla pandemia in questi diciotto mesi è stata improntata, prima dal Governo Conte e successivamente dal Governo Draghi, sulla necessità di modulare le necessarie chiusure, parziali o totali a seconda del momento, e le conseguenti riaperture delle attività commerciali e delle strutture ritenute a forte rischio per possibili contagi

Seguire i dati scientifici, senza fughe in avanti rischiose, e l'avanzare della campagna vaccinale ci permettono oggi di essere in una situazione di vantaggio e di speranza. Somministrare il vaccino a fasce sempre maggiori della popolazione, riuscendo a raggiungere un grado di omogeneizzazione sempre più elevato su tutto il territorio nazionale, è la vera chiave di svolta. Nei momenti in cui si è riusciti a ottenere - pur tra le tante difficoltà e le mille problematiche - un grado di protezione sufficiente, con il conseguente abbassamento drastico degli indici di contagio, è più che mai giusto accelerare, dando finalmente respiro ad attività in notevole sofferenza. È chiaro che, al di là degli aiuti economici, la prospettiva reale di un futuro delineato e ben definito, con punti fermi da cui partire, su cui programmare le scelte di investimento e da cui indirizzare le opzioni di *marketing*, ivi compresi acquisti di materie prime e di logistica, rappresenta la vera ripartenza per le imprese. Tutte le misure previste in questo decreto-legge, che abbracciano anche il nostro vivere sociale, il nostro modo di incontrarsi e di vivere i rapporti interpersonali, rappresentano un segnale forte: finalmente la pandemia è controllabile. Stiamo andando avanti nella battaglia contro il virus. Passano ai nostri occhi - e infondono sicuramente gioia al nostro animo - le immagini dei ristoranti riaperti, dei turisti che ritornano nelle nostre città d'arte e sulle nostre splendide spiagge o dei tifosi che si riappropriano degli stadi fino a pochissimo tempo fa vuoti, così come dei cinema e dei teatri. È importante, però, non far passare il segnale erroneo del «tutti liberi» o dell'«oramai tutto è finito»: sarebbe assolutamente sbagliato perché la gradualità delle riaperture - ripeto giuste e condivise - l'allentamento progressivo delle restrizioni devono e dovranno sempre avvenire nel rispetto delle esigenze di contenimento, nell'applicazione delle misure di protezione individuali e nel controllo rigido e rapido di eventuali nuovi focolai che si potranno verificare ad opera di possibili varianti, quest'ultime sempre in agguato. Abbiamo visto cosa sta accadendo nel Regno Unito. Non bisogna abbassare la guardia. A tal proposito sarebbe indispensabile garantire dosi vaccinali ai Paesi economicamente più deboli, per una questione non solo etica, ma anche sanitaria, per evitare il pericolo del selezionarsi di possibili di possibili varianti, come già successo, d'altronde, che potrebbero diffondersi e - in assenza di una risposta ottimale ai vaccini attualmente disponibili - mettere a rischio il percorso già delineato che ci sta portando realmente fuori dal tunnel. Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto con forza e ripetutamente ai vertici europei l'abolizione temporanea dei brevetti dei vaccini. Il Parlamento europeo ha approvato grazie ai voti decisivi del MoVimento 5 Stelle - un emendamento alla risoluzione sui vaccini, che chiede alla Commissione europea di sostenere la proposta di sospensione temporanea dei brevetti. Il segnale è chiarissimo: da questa pandemia non ci salveremo da soli. Dobbiamo imparare una volta per tutte che siamo tutti sulla stessa barca e che atteggiamenti egoistici potrebbero davvero essere una rovina. Non si può permettere che interessi economici di pochi appartenenti alla ristretta cerchia di *big pharma* prevalgano sulla lotta quotidiana per la vita di centinaia di milioni di esseri umani. Concludo, signor Presidente, con un messaggio di grande speranza, ma, al tempo stesso, di estrema attenzione: riprendiamoci la nostra vita e il nostro futuro, ma avanti adagio. Occorre essere realisti e consequenziali nei provvedimenti, senza demagogia, ma nel solo interesse dei cittadini e a tutela della loro salute psichica e fisica.

improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti

per potersi spostare in entrata e in uscita tra le Regioni, quelle che erano gialle e rosse, anche se adesso ci muoviamo tra quelle gialle e bianche. Diventerà il certificato

e inequivocabile: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, Ancora più importante è il secondo comma, che recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - non porli - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Quindi, nel momento in cui stiamo ponendo tale questione per consentire di spostarsi tra una Regione e un'altra, tra un Paese europeo e un altro, ma anche per partecipare alle feste e ai banchetti di nozze, stiamo facendo qualcosa che va contro questo articolo. Ed è possibile che, in futuro, sia necessario far ricorso a questo certificato anche per presenziare ad altri eventi, come concerti, ai quali adesso è consentito essere soltanto 1.000 all'aperto e 500 al chiuso,

il costo del tampone. Il tampone molecolare, che rimane il *gold standard* per la diagnosi del Covid-19, costa tra i 60 e i 100 euro a seconda delle strutture e delle Regioni. In farmacia costa dai 30 ai 40 euro. E questo per andare ad un concerto e per potersi spostare. Ed è un certificato obbligatorio, per il momento anche a due anni; poi forse diventerà obbligatorio dai sei anni.

«I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.». Diversamente creeremo un Paese per pochi, cittadini di serie A e cittadini di serie B, per andare ad una festa di nozze, ad un concerto, a una manifestazione. Quindi, spero che questa Assemblea

quanto riguarda l'ordine del giorno G8-*bis*.1, il parere è favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti di imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti, nel rispetto dei Regolamenti in materia e delle norme sul *green pass*, la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

favorevole a condizione che, dopo le parole «a valutare l'opportunità», siano inserite le seguenti «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

grazie.

il Governo: a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alle libertà di spostamento

parere favorevole a condizione che, dopo le parole «a valutare l'opportunità», siano inserite le seguenti «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

In apertura della seduta di domani, il Presidente ricorderà la figura di Guglielmo Epifani. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Al termine della commemorazione, si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto finale del decreto-legge riaperture. La seduta sarà quindi sospesa dalle ore 11,45 alle ore 15,30, su richiesta di due Gruppi parlamentari. L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 15,30, prevede il decreto-legge sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e il disegno di legge sulle semplificazioni in materia di procedimenti elettorali, ove conclusi dalle Commissioni. Il calendario dei lavori della settimana comprende inoltre, ove concluso dalla Commissione in sede redigente,

per gli affari regionali e della cultura. Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino. Mercoledì 23, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021. Giovedì 24, alle ore 10, il Ministro della difesa svolgerà un'informativa sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan. Alle ore 15, avrà luogo il *question* *time*. La settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento ai decreti-legge su assegno temporaneo, rafforzamento pubbliche amministrazioni

volevo avvertire l'Assemblea che in Conferenza dei Capigruppo Fratelli d'Italia ha votato contro il calendario di domani. Voglio spiegare le motivazioni per le quali siamo stati costretti a esprimere la nostra contrarietà non sul calendario di questa o della prossima settimana, ma sull'incertezza

d'Italia, tutti dedicati perlopiù al superbonus, con la volontà di migliorare il provvedimento. La maggioranza, così composita ed eterogenea, non trova una quadra

se ci fosse un'avversità esterna; no, l'avversità è interna alla maggioranza, che allora non trova la quadra sui suoi emendamenti, quelli presentati;

che ci verrete a chiedere il voto di fiducia. Vorrei ribadire che tra il Governo Conte e il Governo Draghi andiamo avanti tra procedure d'urgenza, circa 45, e voti di fiducia, circa 13 o 14. Il voto di fiducia è una pietra tombale sui provvedimenti: non consente il dibattito parlamentare, né di migliorare i testi e i provvedimenti, quindi sostanzialmente svuota anche le Aule della loro

questa vostra incertezza e impermanenza e chiede che la Commissione inizi a lavorare sugli emendamenti, che questi vengano analizzati

Senatrice Rauti, la proposta che ha fatto di impegnare i lavori della Commissione non è nella disponibilità dell'Assemblea, quindi non è sottoponibile a un voto.

29 casi di femminicidio in Italia soltanto nel 2021: 29 donne sono state sottratte ai propri cari a causa di compagni o mariti aggressivi, che in molti casi non volevano lasciarle andare e che vivessero libere senza di loro. L'ultimo caso è quello di Alessandra Piga, giovane di venticinque anni, originaria di Maracalagonis, un paese della provincia di Cagliari. A toglierle la vita è stato il suo ex compagno, un ragazzo di origini marocchine, che l'ha uccisa barbaramente sgozzandola, incurante che il figlio e l'amica della vittima fossero in casa. «Dammi l'ultimo abbraccio»: così ha detto Alessandra prima di morire, rivolta al suo ex marito. La donna è stata uccisa al culmine di una lite con un coltello da cucina. Lui, ventinovenne, l'ha uccisa senza pietà. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco, si è fermato il giovane e lo si è arrestato. L'omicidio di Alessandra ci fa pensare alla terribile vicenda di Saman, la giovane diciottenne pakistana che si è scontrata con la ferocia di una cultura retrograda, che tratta le donne come oggetti, prive del diritto di scelta sulla propria vita. Quanto dobbiamo continuare a tollerare culture maschiliste e ignoranti, procreatrici della terribile violenza di genere?

È fondamentale inserire l'aggravante di femminicidio nel codice penale italiano, che già si avvale del codice rosso, un punto di riferimento molto importante nella nostra legislazione. Inoltre, è necessaria una svolta culturale: è di estrema importanza creare nuove professionalità, figure competenti che guidino le famiglie e i giovani, e avviare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di educazione all'interno dei nuclei familiari. Abbiamo bisogno di finanziare un maggior numero di centri antiviolenza, perché ancora insufficienti. Le donne devono sentirsi protette e libere di vivere come credono, e di denunciare, senza temere ripercussioni o peggio, che l'aggressore sia a piede libero dopo pochi mesi di detenzione. È proprio questo fatto che frena e demotiva la vittima, non permettendole di esprimersi: la paura e il terrore che la sua voce non venga ascoltata. signor Presidente, dobbiamo richiedere pene più severe, iniziando dagli abusi domestici: uomini del genere devono essere terrorizzati soltanto all'idea di sollevare un dito contro una donna e devono marcire in prigione, senza se e senza ma.

colleghi, ieri è stata la giornata mondiale dei donatori di sangue. Negli anni abbiamo imparato a riconoscere il valore del dono di sangue, plasma o altri derivati ematici per i pazienti, che grazie a questo gesto di solidarietà possono guarire o, quantomeno, continuare la loro lotta per la vita. Donare sangue è un esempio per i giovani e li educa al rispetto di se stessi, prima ancora che alla generosità verso gli altri, il nostro prossimo cristiano. Ogni singolo donatore ha una sua scala di valori interiore, ma si riconosce comunque in quelli che animano e spingono gli altri a donare. La donazione dev'essere anonima e ci insegna che non esistono pazienti di serie A o di serie B. Il diritto alla salute è universale: non può esserci il «perché lo fai?» o «per chi lo fai?», dove quel «chi» potrebbe essere ognuno di noi o un nostro familiare. Donando sangue si diventa uniti da un filo rosso, che guida il bellissimo viaggio delle sacche donate, scoprire o riscoprire i significati dell'azione solidale, in cui si rinnovano e crescono il senso di appartenenza alla collettività, la volontà di inclusione e di coesione sociale e il senso di responsabilità. Sui valori della donazione del sangue, come sui tanti valori profondi e sentiti del nostro popolo, poggiano le fondamenta della democrazia e della vita stessa della nostra Repubblica. Donare il sangue è donare la vita. *(Applausi)*.

vorrei associarmi alle parole del collega, senatore Mautone, sul tema della donazione di sangue. Questa mattina ho fatto il mio dovere, come tanti parlamentari, perché tra le cose che forse non si conoscono c'è il fatto che, presso la Camera dei deputati, da tempo è in corso un'iniziativa che raduna deputati e senatori, cioè Senato della Repubblica e Camera dei deputati.

C'è bisogno di sangue, in particolare nelle stagioni estive e dopo la vicenda del Covid, e credo che il Parlamento faccia bene non solo a fare un gesto simbolico, che poi è anche effettivo, come la donazione del sangue, ma anche a richiamare le istituzioni e il Governo a una grande campagna di mobilitazione dei cittadini. I cittadini italiani hanno sensibilità e lo hanno dimostrato sul campo: quando ci sono stati appelli delle autorità pubbliche, si sono riversati a donare il sangue e penso ai mesi drammatici che abbiamo vissuto.

con una media di due incidenti mortali ogni ventiquattr'ore. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto oggi ad Avola, in provincia di Siracusa, dove un operaio di quarantacinque anni è morto in un cantiere edile, mentre un suo collega è rimasto ferito dopo il crollo di un ballatoio nel perimetro di un'abitazione privata, dove entrambi stavano lavorando. Due giorni fa si è invece verificato un altro episodio nella stazione ferroviaria di Perugia, in Umbria, dove il capotreno del Frecciarossa per Milano e Torino è stato aggredito da un viaggiatore sprovvisto di biglietto, che gli ha causato la rottura di un braccio: per questo i sindacati del comparto ferrovie hanno indetto per domani uno sciopero di un'ora, per tutto il personale dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, di Italo-NTV e delle società Trenord e Trenitalia, così da portare all'attenzione delle istituzioni i temi della sicurezza sul lavoro. Nel manifestare a nome del MoVimento 5 Stelle e della Commissione lavoro del Senato, che presiedo, la vicinanza personale e istituzionale ai familiari dell'operaio di Avola deceduto oggi e al capotreno vittima dell'aggressione, credo che il Parlamento e il Governo abbiano il dovere di fare di più per affrontare quella che è diventata

Il Paese ha bisogno di una terapia *shock* per ripartire dopo lo tsunami pandemico che, va ricordato, ha visto tanti medici, operai sanitari e infermieri perdere la vita a causa del Covid-19, dopo essersi infettati in reparto o in ambulatorio mentre svolgevano il proprio lavoro. Serve una battaglia di consapevolezza e tocca a noi tutti, alla politica, cominciare a portarla avanti. Partiamo dal lavoro, dalla tutela della vita e della salute. Abbiamo svolto una discussione nel merito per individuare strumenti più idonei a contrastare questa strage silenziosa, cominciando dalle proposte di legge depositate al Senato, come quella del MoVimento 5 Stelle, a firma mia e del collega Romano, per l'istituzione di una procura nazionale del